Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le Commissioni parlamentari bicamerali già convocate in data 25 luglio 2013 - le cui sedute costitutive non si sono svolte - sono nuovamente convocate, per la loro costituzione, domani, giovedì 1° agosto, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo i seguenti orari: - ore 8, Commissione parlamentare questioni regionali e Commissione parlamentare per la semplificazione; ore 14,30, Commissione parlamentare infanzia e adolescenza, Comitato parlamentare Schengen, Commissione parlamentare enti gestori e Commissione parlamentare anagrafe tributaria. Comunico inoltre che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le delegazioni presso le Assemblee parlamentari NATO, Consiglio d'Europa, INCE e OSCE, già convocate in data 25 luglio 2013 - le cui sedute costitutive non si sono svolte - sono nuovamente convocate per la loro costituzione, sempre nella giornata di domani, secondo i seguenti orari: - ore 8, delegazione Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa, presso la sede di Palazzo Valdina, Sala Soprachiesa;

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 10.0.200 (testo 2) e 11.35 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 10.0.200 (testo 2) parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al secondo comma, dopo la parola: "intermedi", delle seguenti: ", nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente,". Il parere sull'emendamento 11.35 (testo 2) è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, alla fine del comma 12-*quinquies*, del seguente periodo: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*bis* e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.". A rettifica del parere precedentemente espresso, formula parere di semplice contrarietà sulla lettera *e)* della proposta 7.800, permanendo parere di nulla osta sulle restanti parti».

regolarmente bollinata senza la nostra condizione, e francamente credo che tali relazioni tecniche - lo dico molto chiaramente - debbano essere viste con maggiore attenzione, perché il principio fondamentale della copertura è quello della contestualità tra l'onere e la copertura. Usare nella relazione tecnica il futuro

Leggiamo con attenzione le relazioni tecniche e nella quasi totalità dei casi siamo d'accordo, ma la responsabilità definitiva è del Parlamento allorquando si esamina il nodo degli oneri e delle coperture. per lo meno su questioni di così grande rilevanza, desidereremmo avere un supporto tecnico assolutamente argomentato e in linea rigorosa con

speriamo di averlo fatto con tutta la precisione e, se necessario, quando rivedremo il provvedimento potremmo addirittura migliorarla, sempre comprendendo fino in fondo qual è lo spirito di questo emendamento, perché forse merita un maggiore approfondimento. Ancora stamattina,

sulla base del quale formulare una decisione che è presa con cognizione piena degli elementi tecnici e della volontà politica: questo è fondamentale per questi grandi emendamenti, così come per i grandi disegni di legge. Pertanto, con la formulazione della condizione abbiamo cercato di riportare la contestualità tra l'onere e la copertura. Lo abbiamo fatto di comune accordo e, come si vede, la relatrice ha accettato la condizione; d'altra parte, ha partecipato ai lavori della Commissione bilancio: ne abbiamo discusso con attenzione, ed è andata bene. Purtuttavia, in questa sede devo ricordare ulteriormente e sottolineare che questa procedura di finanziamento del pagamento dei debiti non è una procedura ordinaria, perché non passa attraverso il bilancio annuale: ciò al fine di incorrere solo molto parzialmente sul *deficit*. Noto che siamo appena usciti dalla procedura per *deficit* eccessivo e tutti insieme desideriamo non rientrarvi. Come è noto, lo sblocco di questi pagamenti, per la per la loro parte capitale, incide sul *deficit;* questo emendamento li esclude: quindi, è coerente con questa impostazione, ma mi pareva giusto sottolinearlo. Anche per i pagamenti di parte corrente, però, c'è una questione europea: non si ha l'autorizzazione ad incidere direttamente sul debito se non È vero che qui, correttamente, al comma 12‑*quinquies*, si richiama la procedura che ci ha autorizzato

da parte del Parlamento, delle grandezze che poi vengono controllate dall'Europa e che sono, in particolare, il *deficit* e poi i saldi che vengono fissati dalla Nota di aggiornamento. Quindi è utile,

che anche per questo emendamento, trattandosi di un pagamento sul debito e non sul *deficit*, è necessario che l'insieme di quella procedura, quando quel Fondo dovrà essere attivato, sia stata messa in opera;

che anche per l'operatività di questo emendamento è necessario l'espletamento di tutta quella procedura che parte dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per arrivare poi a tutte

in Parlamento abbiamo tentato, per un verso, di dare una logica coerenza e, dall'altra parte, di segnare un percorso che si attenga scrupolosamente, trattando di cifre assolutamente rilevanti, alle procedure individuate nel corso delle iniziative legislative.

deve poter operare sulla base di un supporto tecnico rigoroso per effettuare la sua scelta, che poi è tecnica e politica. Se manca uno di questi pilastri, come lei sa, signora Presidente, le cose non vanno bene. E questo a garanzia di tutto il Parlamento e dell'ottimo lavoro che viene fatto in questa sede. *(Applausi

lo Stato sana i suoi debiti nei confronti delle imprese: l'abbiamo fatto con 40 miliardi di emissione di nuovi titoli del debito pubblico, stavamo nei parametri, la procedura sta funzionando, faremo le verifiche con il tempo. In questo caso si agisce sui debiti di parte corrente, quindi non di parte capitale, e non sono una parte esiziale del debito delle pubbliche amministrazioni verso le imprese. Nelle stime della Banca d'Italia sull'ammontare complessivo del debito, che al 15 settembre dovremo avere però certificato da tutte le amministrazioni territoriali e da quelle sanitarie, si parlava di 90 miliardi di euro di *stock* di debito accumulato nei confronti delle imprese. I 40 miliardi che abbiamo messo in campo riducono questo stato di debito. È presumibile che dei 90 miliardi

che non potevamo fare altre manovre analoghe a quelle del decreto paga debiti, abbiamo cercato, con il meticoloso e importante

che richiedono allo Stato il supplemento di intervento per far fronte ai debiti di parte corrente. Si tratta di un'operazione che è stata riposizionata, come ha detto il presidente Azzollini, dal Parlamento.

con aspettativa maggiore al risanamento del rapporto tra amministrazione e imprese, per avvicinarci a quel livello di azzeramento del debito che è auspicabile in ogni Paese civile ed avanzato.

dal Parlamento nel corso di questi mesi, iniziato con il decreto paga debiti e la Commissione speciale per l'esame dei decreti-legge, e che adesso trova una sua applicazione chiamando in causa altri intermediari e prevedendo un meccanismo di garanzia dello Stato nei confronti delle altre amministrazioni attraverso il Fondo

sul controllo della procedura, per verificare che effettivamente questa produca non tutti gli effetti possibili dal punto di vista della corrispondenza burocratica,

stanno arrivando alle amministrazioni e in parte arrivano alle imprese, ma ad un certo punto dovremo sapere - e spero che entro l'anno si possa chiudere questa storia - se abbiamo effettivamente compiuto il passo decisivo per azzerare il debito tra pubblica amministrazione e imprese.

ad esercitare, all'interno di questo testo, tutto quel compito di programmazione economica che la Commissione bilancio ha avuto la possibilità di recuperare. Infatti, al di là delle questioni legate alle opinioni diverse che talvolta emergono tra Ragioneria generale dello Stato e Commissione bilancio, il presidente Azzollini ha specificato e ha sottolineato molto bene prima come questo sia il luogo dell'interpretazione e della mediazione politica nel contesto di un equilibrio di bilancio di cui la Commissione è garante nei confronti di tutta l'Aula. Ma c'è di più.

perché forse non ci consentiranno di raggiungere rapidamente quel risultato. Resta davanti a noi sempre l'esempio del modello spagnolo che in tre mesi è stato in grado di pagare cento miliardi di euro. Ma proprio questo testo può aiutarci a colmare il *gap* e ad aggiungere risorse.

Si completa quindi quel circolo virtuoso che da tempo non si muove più, che da tempo non è più azionato, che fa sì che più sviluppo produca maggiore gettito. Anche attraverso questo strumento possiamo tornare in equilibrio su quella pressione fiscale che quando viene calata su un PIL e un denominatore così basso, come abbiamo sempre detto, determina effetti drammatici

Noi stiamo sostenendo, attraverso questo testo, un'immissione di ricchezza verso le imprese, che tornano in possesso di ciò che avevano anticipato allo Stato, cambiando la loro natura di impresa, visto che si erano trovate a fare da banca allo Stato stesso. Quindi saniamo, al termine di questa difficile procedura, quando arriveremo arriveremo a saldare l'intero debito commerciale della pubblica amministrazione (quantificato, e probabilmente certificato presto, in 92 miliardi di euro), un *vulnus* che non poteva appartenere a un Paese civile e giusto come il nostro. In

poiché ci troviamo in un periodo in cui le imprese sono veramente in sofferenza. Ci sono ancora dei problemi burocratici all'interno delle amministrazioni che non consentono

UPT)-PSI-MAIE)*. Prego, faccio in modo di non essere io di intralcio a chi vuole uscire dall'Aula. signora Presidente. Qualche giorno fa il ministro Giovannini ha ricordato che in Italia ci sono 3 milioni di disoccupati e 2 milioni e 200.000

e nemmeno titolati verso l'occupazione scolastica. La domanda che dobbiamo porci e dobbiamo porre al Governo è se il provvedimento che oggi arriva alla sua votazione finale possa essere considerato sufficiente per dare una risposta

La mia opinione è che debbano essere condivisi i criteri di base (che ricordo: tirocinio, incentivi temporanei alle imprese, trasformazione dei contratti in tempo indeterminato), ma anche che i criteri di base da soli non debbano essere considerati Mi piace vedere alla base di questo provvedimento una rilettura del *welfare* italiano quando si spostano risorse economiche che vengono indirizzate soprattutto verso una una giovane generazione. Noi sappiamo ormai da tempo che le due ragioni di base per le quali l'articolazione sociale ed economica italiana sta venendo meno e crea delle condizioni negative che non favoriscono la crescita e lo sviluppo si ritrovano entrambe alla base di una risposta che questo provvedimento prova a dare. una società decisamente invecchiata (siamo un'Italia rovesciata rispetto a quella degli anni Cinquanta-Sessanta) e le società vecchie non sono in grado di produrre ricchezza, o lo sono con molte più difficoltà rispetto a società che hanno caratteristiche diverse. L'altro fattore è che in Italia non abbiamo più un'organizzazione civica cittadina: quella che è stata la nostra ricchezza nel Medioevo e nel Rinascimento oggi sta diventando il suo contrario. In Italia le città di stampo contemporaneo non esistono più, salvo due eccezioni: Milano per una parte e Roma per l'altra. Se non combiniamo questi due fattori, la mia opinione - e mi rivolgo al Sottosegretario che rappresenta qui il Governo - è che qualsiasi provvedimento rischia di essere zoppicante se non dà una risposta in prospettiva a questa combinazione sinergica di due fattori negativi.

si tengono la mano e non rispondono più a caratteristiche e a condizioni divergenti, perché se non sciogliamo il nodo legato alle questioni sociali, non siamo più in grado di rispondere nemmeno ai diritti civili di base.

Quello che è stato concepito come un registro destinato ai nostri figli è diventato, per metà, un registro cui aderiscono le nostre madri e i nostri padri, perché non è più possibile per chi ha pensioni minime sostenersi per il resto della vita se non ricorrendo a forme di «fidanzamento» (utilizzo questo termine, che può consentire una lettura comune

La quinta e ultima questione ‑ e capisco l'obiezione che potrebbe essere sollevata ‑ riguarda un tema di ordine generale. Capisco che se non c'è sostegno alle piccole e medie imprese italiane, che sono l'articolazione attraverso la quale passa la grande occupazione italiana,

cui ci sono imprese che muoiono per credito anziché imprese che muoiono per debito. Questa è una ragione in più perché venga liquidato, con un'accelerazione, ciò che il Governo, in maniera fruttuosa, ha previsto Una questione finale, signora Presidente, e ho concluso. Ci sono tre fattori, accanto ai due che ho citato all'inizio, che persistono un'alta sperequazione tra i redditi, una bassissima mobilità sociale e l'allargamento della fragilità della base sociale del Paese. Appartengo ad una categoria che sostiene ancora oggi vigente e vivente la differenza fra destra e sinistra. Anzi, c'è un punto che sottolinea tale differenza, ed è la redistribuzione della ricchezza. Siamo di fronte a un Governo che combina la destra e la sinistra, e mi fa piacere pensare che entrambe le squadre giochino nella stessa metà del campo;

rappresentante del Governo, in questo momento in Italia si intrecciano almeno tre problematiche di natura economica e finanziaria che impattano sui nostri conti pubblici e sul contesto politico, essendo diretta derivazione dei programmi elettorali delle forze politiche che sostengono il Governo, e sono le imposte sulla casa, le imposte sui consumi e quelle sul lavoro.

di interventi per dare una scossa forte alla ripresa economica di cui ha bisogno il Paese. Ancora una volta, oggi siamo chiamati - e noi sosteniamo questo cammino - ad assumere decisioni che hanno la forma e la sostanza del tampone rispetto a problematiche che vive il nostro Paese. Debbo dire che anche dal dibattito parlamentare pare essere emersa questa consapevolezza,

stiamo discutendo di una crisi terribile, profonda, che ormai da anni si registra nel nostro Paese, ma che in maniera più forte, decisa e pesante vive il 50 per cento del territorio del nostro Paese

motore produttivo della nostra Europa, anziché partecipare alla competizione mondiale per la ricerca di nuovi continenti, come stanno facendo gli Stati Uniti da un lato e i colossi del Sud-Est asiatico dall'altro, aggredendo il continente africano come nuovo campo di produzione, sviluppo e vendita dei propri prodotti, ha scelto la strada più semplice, che è quella di aggredire i propri alleati europei e fare politiche che le hanno consentito e che vorrebbe le consentissero ancora di di conquistare i nostri mercati e la nostra capacità produttiva. Questo è il momento che stiamo vivendo. Non è una lotta tra Nord e Sud e tra Sud e Nord. È una lotta del sistema Paese e del sistema Italia, che se non è competitivo nel suo insieme sarà debole e non riuscirà a superare questa sfida. Ma io voglio argomentare. Debbo dire che

ci si attende da questo rapporto qualcosa che possa essere indicativo ed una traccia rispetto allo sviluppo che ci si aspetta. Mi limiterò a leggervi soltanto i titoli dei paragrafi e lascio alla vostra immaginazione capire ciò che si nasconde dietro i titoli dei paragrafi. «2012-2013: ancora in crisi l'area dell'euro». Punto 2: «L'Italia risente di più dell'esaurirsi della fase di ripresa». 3: «Dopo la mancata ripresa nel 2010-2011, il Sud in più forte recessione nel 2012». «Si consuma sempre meno e non si investe più». Punto 5: «Tutti i settori coinvolti dalla crisi». Punto 6: «L'andamento delle Regioni italiane» (dove troverete le previsioni di sviluppo sono in una media nazionale dello 0,8, ma questo 0,8 è composto dallo 0,9 delle Regioni del Centro Nord e dallo 0,1 delle Regioni del Centro-Sud). «Le aree deboli dell'Europa maggiormente colpite dalla crisi» (e vi troverete enumerate soprattutto le Regioni del Mezzogiorno). Punto 8: «Industria del Sud: investimenti crollati di quasi il 50%. 9: «Il lavoro è sempre più un miraggio». Punto 10: «Dualismo territoriale e dualismo generazionale». Punto 11: «1.850 mila giovani NEET nel Mezzogiorno, lo spreco dei cervelli». Punto 12: «L'emergenza femminile».

«Un terzo delle famiglie meridionali a rischio povertà». Questo è il rapporto della SVIMEZ. Questo è uno strumento di lavoro che non vorremmo utilizzare perché, naturalmente, il nostro compito è quello di creare speranza e prospettive. Dobbiamo partire però da questa situazione di fatto. Per fare questo, signor rappresentante del Governo, abbiamo bisogno di progetti organici di sviluppo. Abbiamo bisogno di inquadrare questi problemi nell'ambito di un'azione complessiva di governo. Non vorremmo più vedere in quest'Aula provvedimenti tampone, che sono pur necessari, ma solo se inseriti nel quadro di una complessiva prospettiva di crescita. Le voglio comunicare un dato che mi angoscia. La regione Sicilia, che ha più di 5 milioni di abitanti, in una proiezione per il 2050 vedrà calare la propria popolazione di un quarto e il proprio PIL di un terzo.

tutti i Paesi del Nord Africa, che si affacciano sullo stesso mare, avranno una media di età di 25 anni nel 2050. 2050. Questi non sono i problemi, cari amici della Lega, del Sud che chiede e del Nord che ritiene che si è troppo dato e che non bisogna più dare: è un problema di sistema Italia. È un problema complessivo di crescita. Rispetto a questo problema, avete visto che tipo di provvedimento è stato messo in campo? Signor rappresentante del Governo, noi lo voteremo perché abbiamo dato fiducia e diamo ancora fiducia e credito a questo Governo, ma è previsto che possano avere agevolazioni per il lavoro dei giovani che non abbiano più di 29 anni, giovani che non abbiano frequentato la scuola dell'obbligo, ovvero che si sono fermati alla terza media.

non può aiutare il Paese nell'aumento del PIL e della produzione. È un Mezzogiorno che vi trovereste eventualmente tanto più in casa dalle vostre parti. Siccome da talune espressioni avvertiamo che non vi fa particolarmente piacere, evitiamo e votate anche voi, amici della Lega,

Presidente, la nostra dichiarazione di voto parte con un rammarico perché avremmo voluto votare a favore di un provvedimento che ha come obiettivo principale l'affrontare il problema della disoccupazione giovanile e della disoccupazione in genere. Avremmo voluto farlo e forse l'avremmo fatto se questo provvedimento non fosse stato, nel merito, espressione diretta di una vecchia filosofia e, soprattutto, di un approccio monoculturale. Interviene, tentare di rilanciare l'occupazione attraverso forme di aiuto alle imprese e attraverso un'ulteriore flessibilizzazione

nell'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento che, come è noto in letteratura, sono indicati come strumenti a favore del tirocinante e devono costituire

a costo inferiore, con l'intervento di manodopera a basso costo.

della rappresentanza sindacale e si riduce la possibilità positiva delle relazioni sindacali rispetto agli obiettivi comuni di rilancio dell'economia e della capacità produttiva di questo Paese. Avremmo voluto votare a favore, ma per queste ragioni non lo faremo. Avremmo voluto votare a favore, come abbiamo votato a favore di molti articoli, non ultimo quello sui debiti della pubblica amministrazione, che abbiamo discusso in Commissione bilancio e approfondito nelle altre Commissioni di merito, oppure come abbiamo fatto per la flessibilizzazione dei contratti del settore turistico o per altri articoli che pure sono meritevoli di attenzione, articoli che riguardano l'inserimento lavorativo di soggetti che subiscono, purtroppo, una condizione di disabilità.

frutto più di ambienti burocratici, un po' fuori dalla considerazione diretta dei problemi del Paese per cui sono più studiate a tavolino che nella relazione diretta con il problema, con il bisogno;

per cui in questa sottospecie di provvedimenti normativi «a minestrone» capita che qualcosa non sia da considerare perché estranea ad una materia senza che questi provvedimenti abbiano ad oggetto una materia, giacché ne contengano 10, 12, 15 di materie. provvedimento è ancora peggio rispetto a questo: Quello «del fare» non è un minestrone, è di più.

si è registrata una frattura che va sanata. Lo dico soprattutto nell'interesse del centrosinistra nel suo complesso e in modo particolare del Partito Democratico, che noi non vogliamo sia il nostro alleato

confronto che si attiva tra schieramenti che hanno opinioni, culture, visioni, prospettive diverse; e voi rinunciate alla vostra: infatti, in questo provvedimento - badate - rinunciate alla vostra, c'è solo qualche rimasuglio,

Ed è questa la ragione: non sono le vicende di questo o quell'altro personaggio politico, per quanto importante. È la ragione della vostra rinuncia a rappresentare in questo Paese i valori della sinistra, primo fra tutti il lavoro, perché questo provvedimento è un aiuto all'impresa,

al problema. Infatti, tra l'uovo e la gallina io sono convinto che nasca prima l'uovo; e siccome sono convinto che nasca prima l'uovo, nessuno mi può togliere dalla testa che è il lavoro che fa l'impresa e non il contrario, perché è l'applicazione della volontà e della competenza che ha costruito settori produttivi importanti in questo Paese.

per salvare insieme a noi la prospettiva di questo Paese di organizzare uno sviluppo duraturo, in un ambiente democratico,

Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, a distanza di una settimana ci ritroviamo in quest'Aula ad esprimere il nostro voto su un decreto-legge recante misure in favore di famiglie e lavoratori. Nuovamente un decreto-legge, nuovamente l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte del Governo. Signori del Governo, voi non siete i professorini guidati da Monti che tutto potevano, che erano al di sopra di ogni regola, al di sopra della Costituzione, che erano stati chiamati dall'alto e non votati dal popolo per fare il gioco sporco. Caro presidente Letta e vice presidente Alfano, voi avete una responsabilità politica una maggioranza ampia che vi sostiene, non perché non c'è alternativa ma per scelta, e non avete il riconoscimento internazionale dato per dato ma ve lo dovete meritare. Quindi, signori del Governo, vi chiediamo di abbandonare i sistemi da *soviet*, di iniziare a confrontarvi con il Parlamento, di entrare nel merito delle misure che volete varare con il coraggio che deve contraddistinguere un Governo politico. Monti è stato condannato, non certo dalla storia (troppo per un Presidente del Consiglio di un Governo così mediocre), ma dal popolo e dai numeri; numeri che dimostrano palesemente, da un lato, i conti in peggioramento e, dall'altro, l'aumento esponenziale della disoccupazione, in uno scenario di forte depressione e recessione! Presidente del Consiglio, lei è alla guida di una maggioranza che, seppur variopinta ed originale, rappresenta il popolo, rappresenta i cittadini che con il loro voto hanno voluto fortemente voluto - un Governo a guida politica dopo la pessima esperienza dei tecnici. Basta rinviare, non decidere, posticipare, allungare i tempi. È ora che il suo Governo faccia una scelta chiara: o vive o muore. Non può più sopravvivere; una linea politica e programmatica la dovete decidere. Noi della Lega siamo all'opposizione, ma vogliamo fare un'opposizione seria e responsabile. Noi della Lega non vogliamo fare un'opposizione fine a sé stessa; non vogliamo aprire il Parlamento con un apriscatole. Vogliamo far uscire il Paese dalla crisi; vogliamo dare una speranza ai giovani che cercano lavoro, che vogliono sposarsi, che vogliono mettere su famiglia. LN-Aut).*Vogliamo un Nord che sia protagonista del cambiamento di questa Europa tecnocratica. Vogliamo andare verso un'Europa nuova, un'Europa dei popoli, non unita soltanto ed unicamente dalla stessa divisa monetaria e non basata unicamente su una partecipazione a quote. Sogniamo, vogliamo un'Europa politica capace di tutelare le differenze dei cento popoli che la compongono; un'Europa che sappia essere protagonista delle politiche mondiali. Il decreto-legge su IMU e cassa in deroga si è rivelato una farsa, considerato che non si è affrontato il problema, bensì lo si è solo rinviato nel tempo, tant'è che la stessa compagine governativa lo aveva definito un decreto-ponte. Parimenti, anche questo suona a noi come una beffa. Ma per quanto tempo credete di riuscire a prendere in giro i cittadini? Se solo una volta vi degnaste di fare un giro in mezzo alla gente! Provate a scendere dall'auto blu e a muovervi senza scorta tra i cittadini, tra coloro che ci hanno eletto (e permettemi di ricordare che sono loro che ci stanno pagando lo stipendio), e subito vi renderete conto che non sono ignoranti come voi credete! I cittadini sono ben informati e sanno bene che questo Governo non è in grado di fare niente; non è in grado di prendere una decisione, ma è bravissimo a rimandare. Sull'IVA è stata presa, come per l'IMU, una decisione artificiosa. Tutti sappiamo che l'aumento dell'IVA causerebbe un minor gettito, con ovvia conseguenza di maggiori difficoltà per le imprese. Rimandate l'aumento di una tassa, per aumentarne un'altra nell'immediato per avere la copertura (vedi IRPEF ed IRAP). Non vi vergognate nel proporre queste soluzioni? Tante parole, tante promesse, ma nessuna decisione tranne quella di aumentare le tasse. State giocando con la vita ed il futuro dei cittadini. Secondo voi, queste decisioni sono in linea con i tanto decantati intenti di voler sostenere la ripresa economica delle imprese? Così pensate di rilanciare il Paese Italia? Così credete di favorire la crescita occupazionale? Se continuate così la stabilità del Paese corre forti rischi. Voi vi preoccupate della stabilità dei conti, di rimanere entro i parametri europei, mentre dovreste preoccuparvi della stabilità del nostro Paese. Quando un popolo è alla fame, per quanto sia civile e democratico, può avere delle reazioni incontenibili. Un'altra cosa è veramente vergognosa: usare due pesi e due misure nei confronti dei cittadini del Nord e del Sud. Io parlo da donna del Nord che, fino a qualche giorno prima della sua elezione, lavorava in una fabbrica, e le mie amicizie, ancora oggi, sono con chi ha trascorso la sua vita all'interno della fabbrica insieme a me. Quando incontro i miei amici, oltre che lamentarsi, mi chiedono: «Perché mio figlio che è nato al Nord è trattato diversamente da un ragazzo nato al Sud?». Cosa devo rispondere alla mia gente quando mi chiede: «Perché al Sud ci sono incentivi e detassazioni per i nuovi assunti e al Nord no?». Cosa devo rispondere? Devo rispondere che, dopo aver passato una vita di lavoro, di sacrifici e di tasse pagate per aiutare il Sud, per l'ennesima volta al Nord ti devi arrangiare e al Sud ci pensa lo Stato? Vi posso dimostrare con dati alla mano che, come per il decreto cosiddetto IMU-cassa in deroga, il varo di questo provvedimento è stato accompagnato da eclatanti annunci e proclami, come quello del presidente Letta che, nel comunicare l'eventuale arrivo dall'Europa di 1,5 miliardi dì euro per il lavoro, affermò: «Ora le imprese non hanno più alibi per non assumere». Il Ministero del lavoro, in una nota rilasciata giorni fa, riconosce che questo decreto rappresenta solo un primo passo della strategia del Governo, perché le vere e concrete misure saranno definite soltanto dopo che le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la «Garanzia giovani». Anche questa volta stiamo per licenziare un provvedimento che, nel concreto, non serve al rilancio occupazionale, perché reca interventi parziali e limitati, privi di prospettive di lungo periodo, e misure eterogenee carenti di una progettualità complessiva. Dei tanti obiettivi dichiarati (promozione dell'occupazione, incentivi per i giovani, interventi in favore della coesione sociale, eccetera), quello che attua questo provvedimento è l'ennesimo assistenzialismo nei riguardi dei disoccupati ed inoccupati del Sud, finendo per sussidiare attraverso la decontribuzione l'assunzione di giovani residenti nel Mezzogiorno. Non è vero che le Regioni del Mezzogiorno sono molto povere, con forti carenze di posti di lavoro e pertanto necessitano di particolare attenzione. Non è possibile né accettabile che, in nome di una perdurante questione meridionale, si continui a sprecare risorse e denaro a danno di quelle Regioni che rappresentano il traino dell'economia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo* *LN-Aut).* Voglio ricordare un'indagine del centro studi Datagiovani, condotta incrociando i dati AIRE con quelli dell'ISTAT sulla disoccupazione negli ultimi cinque anni, cioè gli anni di maggiore crisi. Tale indagine, prendendo in considerazione l'incremento percentuale della disoccupazione Regione per Regione, ha concluso che le sofferenze maggiori si sono avute nelle zone settentrionali del Paese, con in testa l'Emilia-Romagna dove i disoccupati sono più che raddoppiati passando da circa 65.000 a 150.000, ed in Lombardia dove da 168.000 disoccupati del 2008 si è passati a oltre 346.000 nel 2012. Questa ricerca conferma un comportamento dei giovani rispetto al lavoro già comunemente noto, e cioè che mentre i giovani del Nord sono pronti ad emigrare pur di cercare un'occupazione, nel Sud preferiscono restare assistiti e sussidiati a casa propria.

contrariamente al Mezzogiorno ove la crescita dell'emigrazione si attesta intorno al 13 per cento. Riporto questi dati e questa ricerca per invitare il Governo ad avere anche un'altra visione delle cose, a guardare l'emergenza occupazione e la disoccupazione giovanile anche da un'altra prospettiva, perché le politiche di penalizzare il laborioso per sostenere il bisognoso non portano ad alcunché. In conclusione, ripeto un'altra frase che sento spesso tra la mia gente del Nord e che rende benissimo l'idea dello stato d'animo in cui sta vivendo un popolo. In lingua veneta si dice: «A semo becchi e bastonà». Questa frase, tradotta, significa: oltre il danno, anche la beffa. Siete solo capaci di prendere in giro gli italiani e, in particolar modo, il Nord. Per questi motivi, esprimo, a nome del Gruppo della Lega Nord e Autonomie, che rappresento, il voto contrario al provvedimento, ricordando al Governo che la fiducia va conquistata e che per guadagnarla bisogna passare dalle parole ai fatti.

consapevole, tuttavia, che esso non sarà, ancora una volta, risolutivo, né capace di affrontare i nodi strutturali sulle due tematiche che sono oggetto del decreto-legge. Mi riferisco alle due tematiche prevalenti: quella del lavoro (in particolare del lavoro giovanile) e quella della pressione fiscale. Naturalmente non sottovalutiamo assolutamente anche il valore simbolico di questo provvedimento, che è stato adottato dal Governo Letta subito dopo un importante Consiglio europeo in cui c'è stato un protagonismo italiano interamente focalizzato sulla questione del lavoro giovanile, che è diventato uno dei punti centrali dell'agenda. questo sia un passaggio molto significativo della prospettiva e del lavoro dell'Europa, nonché di quella che sarà l'impostazione dell'agenda europea nel semestre italiano, che è in corso di preparazione. Tuttavia, dobbiamo sottolineare, ancora una volta, che i caratteri strutturali di questo tema non sono ancora minimamente sfiorati. Sicuramente ci sarà un beneficio per l'incentivo che viene dato ai datori di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, ma non sarà il beneficio di diciotto mesi a cambiare ciò che oggi condiziona il mercato del lavoro e lo rende quanto mai incerto: mi riferisco alla precarietà delle prospettive, che induce i datori di lavoro a non assumere giovani in assenza di una dinamica dell'economia che prometta crescita in modo stabile, nonché al dualismo del mercato del lavoro, dal punto di vista sia del costo delle diverse forme contrattuali

disponibile ad avviare almeno una sperimentazione di forme nuove che consentano una diversa e più semplice modalità di separazione

Credo che sulla formazione professionale occorra realizzare una rivoluzione profonda e affrontare con le Regioni un discorso di chiarezza, perché credo che uno dei maggiori *deficit* del nostro mercato del lavoro

sottratta anche alle linee guida strategiche dello Stato, devoluta alla competenza delle Regioni e a gestioni quanto più opache possibile. Abbiamo fatto un piccolo confronto con il Governo sull'esigenza di analizzare fino in fondo i risultati delle politiche pubbliche in materia di formazione professionale. Credo che questa sia una necessità assoluta per riorientare i giovani verso sbocchi realmente produttivi. Ovviamente, però, ciò che occorre fare è rimettere in moto l'economia, far riavviare la crescita e rendere più dinamico un mercato che oggi appare quanto mai asfittico. Non sono misure di carattere strutturale questo ci preoccupa molto. Noi vogliamo incalzare il Governo su questo aspetto perché tutte le riforme che possono aiutare ad agganciare la crescita devono intervenire presto, altrimenti questo spiraglio, che anche il ministro Saccomanni ha dichiarato di intravedere all'orizzonte, rischierà di non essere a beneficio della nostra economia o di esserlo troppo poco, e rischiamo di riprodurre quello che già in passato si è realizzato, cioè amplificare, proprio nei momenti di crescita, la distanza tra noi e altri Paesi europei. Per questo, anche il rinvio a settembre, che è stato citato, deciso dal ministro Giovannini del confronto con le parti sociali proprio sul mercato del lavoro ci preoccupa, perché non vorremmo che questo fosse l'inizio di una progressiva dilatazione che appunto accentuerebbe questa tendenza al rinvio che ci sembra preoccupante, perché vediamo che il fattore tempo - un fattore purtroppo ignorato nella storia italiana, per cui riforme indispensabili vengono rinviate per vent'anni - possa essere trascurato anche nell'azione di questo Governo. L'altro punto toccato dal decreto è quello del rinvio dell'aumento dell'aumento di un punto dell'IVA, la cui storia noi conosciamo bene: dipendeva da una copertura insostenibile decisa dal Governo Berlusconi-Tremonti. Si è deciso di sospenderla fino a novembre, ma anche in caso consapevoli delle difficoltà di bilancio che, una volta che si vanno a vedere i numeri, diventano molto stringenti e quindi tutte le posizioni retoriche svaniscono.

tuttavia su imprese che soffrono per mancanza di liquidità anche questo aumento di acconto può determinare un effetto depressivo da una parte sul reddito delle persone fisiche e dall'altro sull'attività economica delle aziende, ma soprattutto si dà il segno che sempre lì si va a pescare, cioè che non vi è uno sforzo di compensare le minori entrate con minori spese. L'ultimo esempio più eclatante è proprio in questo decreto, all'articolo 11, dove si autorizza la Regione Trentino-Alto Adige, che credo di risorse e di entrate fiscali non manchi, ad aumentare l'addizionale IRPEF per coprire il pagamento dei debiti dell'amministrazione. Trovo questo veramente inaccettabile, perché se la Regione Trentino-Alto Adige, che è la più ricca e ha una distanza tra fabbisogni ed entrate, non riesce a diminuire le spese per pagare i debiti, credo che questo non possa essere un metodo di lavoro. Questa è una norma che è stata inserita, forse poco notata, ma a mio avviso indice di un approccio culturale che non non possiamo accettare. Siamo in verità consolati, nell'approvare questo provvedimento, dall'inserimento dell'emendamento 11.35 (testo 3), che oggi il Senato ha approvato, un emendamento importantissimo, su cui si è lavorato per mesi, che va nel senso di agevolare la liquidazione dei dei debiti delle pubbliche amministrazioni assistendoli con una garanzia dello Stato e quindi incidendo molto poco sul *deficit* e sul debito, ma aumentando la liquidità che può andare nel sistema, e che credo sarà la vera manovra di politica economica che può ridare fiato all'economia nei prossimi mesi. Quindi, la speranza è che non ci siano ritardi burocratici.

Quindi credo che vada molto valorizzata la decisione presa oggi, in quanto è un passaggio significativo che può dare, questo sì, un orizzonte alle imprese, che vedono la possibilità possibilità di acquisire liquidità ma anche di sbloccare maggiore disponibilità delle banche al credito. Infatti, è chiaro che i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato riducono i *ratio* patrimoniali a cui sono tenute le banche e quindi reimmettono capacità di credito nel sistema. Ci auguriamo che con il lavoro che stiamo facendo in Parlamento e con il pungolo che noi continueremo a rappresentare nei confronti del Governo, nei prossimi mesi si potrà continuare nell'opera di riforme strutturali di cui abbiamo assoluta urgenza.

ad una persona che muore di sete non si può dare l'acqua con il contagocce. Le misure previste nel decreto che ci troviamo a discutere sono dei piccoli rattoppi alla disastrosa situazione del mercato del lavoro in Italia. Questi interventi, seppur in taluni casi condivisibili, non avranno rilevanza nel lungo periodo e sono proprio gli interventi di lungo periodo ad essere improrogabili e necessari. Le cifre parlano chiaro: dall'ultimo rapporto ISTAT, il tasso di disoccupazione si attesta al 12,2 per cento; oltre 6 milioni di italiani sono cittadini inoccupati o disoccupati. In Italia si trova un terzo degli 8,8 milioni di individui (in maggioranza donne) che nei Paesi dell'Unione europea dichiarano di non cercare lavoro. Ben 2 milioni di questi individui sono cittadini tra i 30 e i 54 anni. Ai 6 milioni di senza lavoro vanno sommati tutti i cittadini che, pur percependo una retribuzione, vivono al di sotto della soglia di povertà. Sono 172.000 i posti a rischio nelle piccole e medie imprese, migliaia gli operai a rischio di perdita del posto di lavoro, centinaia le aziende in crisi industriale. Il sistema produttivo italiano si impoverisce, le aziende chiudono, vengono delocalizzate o vendute. Come vogliamo affrontare questa crisi? In che modo l'Italia può affrontare la crisi dovuta alla globalizzazione? Come può mantenere la propria identità culturale, sociale e politica? L'Europa ci impone misure per il contrasto della disoccupazione giovanile: che ben vengano, ma, visto l'altissimo tasso di disoccupazione, il Movimento 5 Stelle si chiede quali motivazioni abbiano condotto questo Governo, quelli precedenti e i parlamentari italiani eletti in Europa a non chiedere la previsione di misure a contrasto della disoccupazione che ha colpito e colpisce non solo i giovani, ma tutti i cittadini italiani, in special modo la fascia d'età compresa fra i 30 e i 54 anni. Non si può e non si deve far credere di voler incrementare le prospettive occupazionali, peraltro proponendole come soluzione alla crisi, impiegando esclusivamente le uniche risorse che l'Europa ci ha concesso. La direttiva europea ci impone la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, azione assolutamente necessaria per porre fine alla frammentazione degli stessi, frammentazione degli stessi, messa in atto - ricordo - dalle innumerevoli norme che negli ultimi anni si sono susseguite, ciascuna a tutela degli interessi dei singoli e certamente non a tutela del cittadino inerme. Non abbiamo bisogno di due anni per riorganizzare tutto, lo si può fare anche in un anno. Riorganizzare vuol dire anche monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza di quanto fino ad oggi implementato; analizzando i punti di forza e i punti di debolezza, si può ricostruire e ripensare un sistema di *welfare* più efficiente. Ma se a valutare sono gli stessi attori che ne hanno provocato la frammentazione, ci domandiamo a cosa porterà tutto questo. I programmi di politica attiva del lavoro messi in atto e affidati agli innumerevoli enti figli della frammentazione dei servizi per l'impiego quali risultati hanno conseguito? Se alla luce di tale valutazione i risultati sono stati al di sotto di quanto richiesto, noi del Movimento 5 Stelle ci chiediamo quali motivazioni spingono il Governo a mantenere tali costosi apparati. Nel portale «Cliclavoro», attivo dall'ottobre 2010, sono registrati ad oggi meno di 400.000 *curriculum*. Le statistiche dicono che solo il 7 per cento dei soggetti registrati ha ricevuto un'offerta di lavoro. Questo dato è sufficiente per far comprendere che vi è stato un problema non solo nella diffusione del portale, ma anche nella progettazione informatica e gestionale dello stesso. Quante risorse sono state impiegate per lo sviluppo, la conduzione, l'aggiornamento e la diffusione del portale in questi ultimi tre anni? Il parere del Movimento 5 Stelle sull'implementazione della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro è positivo. Il Governo però si impegni a mantenere quanto enunciato e legiferato, partendo innanzitutto dalla valutazione di quanto fino ad oggi attivato e correggendo i precedenti errori, in modo che la creazione della banca dati unica costituisca il primo passo per una riforma strutturale del *welfare*. Riguardo al contratto di apprendistato, ci domandiamo: perché togliere forza allo stesso inserendo gli incentivi di cui al comma 2 del decreto? Perché non dedicare invece quegli incentivi alla fascia di età compresa tra i 29 e i 35 anni, Per quanto inerente all'articolo 7 del decreto, risulta distruttiva, a livello ordinamentale, la previsione con cui si può assumere a tempo determinato senza alcuna specificazione delle ragioni che determinerebbero la temporaneità della prestazione, con ciò violando quanto statuito dal legislatore europeo. Il decreto inoltre prevede che la pubblica amministrazione possa dare in appalto a cooperative un determinato servizio senza incorrere nell'obbligo da parte della stessa pubblica amministrazione di retribuire i lavoratori interessati in caso di inadempimenti dell'appaltatore. Questi sono alcuni degli esempi attraverso cui il Governo intende aiutare le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno si affannano nella ricerca spasmodica di un reddito che consenta loro un accenno di vita libera e dignitosa, come sembrerebbe statuire l'articolo 36 della Costituzione. Ancora una volta, le scelte del Governo, così come quelle dei suoi predecessori, sono rivolte a creare, anzi, a consolidare, l'esistenza dì una classe di lavoratori poveri e senza diritti, con ciò tradendo i principi sanciti nella nostra Costituzione, in particolare dall'articolo 4, secondo cui la funzione che il lavoro deve svolgere nella società è quello di mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona, e non di merce necessaria alla massimizzazione dei profitti Il lavoro è da intendersi quale strumento personale di realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta. In tal senso, la libertà di scelta del lavoro diventa bene comune. Non c'è più tempo. Gli italiani muoiono di fame, l'economia sta facendo passi indietro, le aziende chiudono, gli imprenditori si uccidono, le speranze e il futuro dell'Italia sono quasi nulle. È arrivato il momento di agire, con coraggio, con la forza che viene dal grido di aiuto delle famiglie, degli imprenditori e dei bambini senza futuro. Un'economia sana si fonda su principi razionali, ma soprattutto lungimiranti. È necessario riconoscere il male che attanaglia l'Italia e combatterlo con forza. Non possiamo pensare che dei piccoli interventi possano cambiare lo stato di emergenza in cui il nostro Paese si trova. Non svendiamo la nostra Nazione e il suo patrimonio. Non buttiamo via i sacrifici dei nostri genitori e dei nostri nonni. Non guardiamo agli interessi dei singoli. Osserviamo l'Italia dal punto di vista di tutti i cittadini italiani, perché quei cittadini siamo noi! Noi in quest'Aula li rappresentiamo tutti e ognuno di noi è portavoce del malessere del nostro Paese. Ecco, occorre prendere alla lettera il nostro ruolo. È necessario che ognuno di noi senta sulle proprie spalle, lo dico ai colleghi,

non trova lavoro malgrado il suo *master*, il problema è nostro, perché Mario è nostro fratello. Se Giovanni, imprenditore quarantacinquenne, è costretto a chiudere la sua impresa, il problema è nostro, perché Giovanni è nostro fratello. Se Anna è costretta a chiudere la sua azienda tessile e mandare a casa i suoi venti impiegati, il problema è nostro, perché loro sono la nostra famiglia. Se Paolo si trova in una situazione di disagio sociale, se la sua azienda è in crisi e lui e i suoi colleghi sono in cassa integrazione senza prospettive di rientro, il problema è nostro, perché anche loro sono nostri fratelli. Se Giovanni, Paolo e Francesco si uccidono perché attanagliati dai debiti e disperati, signori, il problema è nostro. Per tali ragioni, il Movimento 5 Stelle ritiene che si debbano attuare misure immediate a contrasto della povertà che riportino dignità alla famiglia, al cittadino, alle imprese e all'Italia: riforma del *welfare*; riduzione delle retribuzioni e delle pensioni d'oro; redistribuzione della ricchezza; una seria lotta all'evasione fiscale; incentivi alle aziende italiane (ripeto: italiane), non "Piano destinazione Italia", non vendita dei marchi italiani alle aziende estere, non "Piano devasta Italia"; riduzione dell'orario di lavoro (lavoriamo tutti e facciamo in modo che ciascuno si senta parte integrante della società); immediata istituzione del reddito di cittadinanza. Mi rivolgo... PRESIDENTE. Ha esaurito il tempo a sua

Signor Presidente, il Gruppo del PdL voterà a favore di questo provvedimento, che risponde all'emergenza determinata da un mercato del lavoro che, nell'ultimo anno, ha registrato il peggiore declino nell'area dei Paesi industrializzati. Siamo stati uno dei Paesi in ambito UE e OCSE che aveva saputo contenere l'impatto della grande crisi sul mercato del lavoro grazie al massivo impiego di ammortizzatori sociali dedicati alla continuità dei rapporti di lavoro e alla vigenza della legge Biagi con le sue diffuse flessibilità regolatorie. Poi, in un contesto ancor più deteriorato dal prolungarsi della crisi, l'alto costo indiretto del lavoro e le molte rigidità normative, le persistenti insufficienze del sistema educativo e formativo hanno congiurato contro l'occupazione. Per queste ragioni una compiuta risposta all'emergenza occupazionale dovrebbe realizzarsi in termini di meno tasse, meno regole, più competenze. Il Governo ha avviato un'azione di contenimento del costo indiretto del lavoro azzerando i contributi relativi a un determinato volume di contratti permanenti per i giovani fino a trent'anni. Essa è parte della più ampia proposta che avevamo presentato nel corso del confronto elettorale, e come tale la condividiamo e la votiamo. Desideriamo però una coraggiosa azione rivolta a semplificare sensibilmente la complessa disciplina introdotta dalla legge Fornero abbiamo proposto di ancorare questa deregolazione all'autentica opportunità offerta dall'Esposizione universale di Milano. Nei tre anni che ci separano dal compimento degli eventi che la realizzano potremmo mobilitare diffusamente le energie della Nazione nella prospettiva degli straordinari flussi turistici attesi e della vetrina globale che oggettivamente si determinerà. Come hanno concordemente osservato le massime cariche dello Stato e del Governo, l'Expo può rappresentare per un Paese depresso ed affetto da processi di disgregazione l'occasione di rovesciare il circolo vizioso, una sorta di catalizzatore della voglia di riscatto che rimane soprattutto in coloro che conservano l'attitudine a rischiare e ad intraprendere o nei molti giovani che possono cogliere questo appuntamento per risolversi a fare ciò che ancora considerano con incertezza. Insistiamo quindi a chiedere norme più agevoli per i contratti a termine e per l'apprendistato, la cui formazione aziendale rimane di incerta definizione e certificazione, regole più consone ai progetti di ricerca, alla cui temporalità devono correlarsi le tipologie contrattuali, il ritorno alla legge Biagi per il lavoro intermittente, per l'uso diffuso dei *voucher*, specie in agricoltura e nei servizi, e per le collaborazioni a progetto. Possiamo fare lavoro non solo nelle manifatture ma anche nel turismo, in agricoltura, nei servizi alla persona e nell'industria culturale. E non basta il rinvio alle parti sociali, che a legislazione vigente possono fare ben poco, come si è visto nell'accordo intervenuto tra sindacati e Expo Spa. Confidiamo pertanto che, ove le parti sociali non addivenissero alla condivisione di modifiche, anche sperimentali e transitorie, alla legge Fornero, il Governo non si sottrarrà al dovere di proporre al Parlamento misure utili a incoraggiare, a intraprendere e ad assumere, impegnando la maggioranza a sostenerle oltre ogni contrapposizione ideologica. Così come auspichiamo che si svilupperanno, anche attraverso la leale collaborazione tra Stato e Regioni, le azioni rivolte a rafforzare l'occupabilità delle persone, a partire dai più giovani, favorendo quanto più possibile l'integrazione tra scuola e lavoro, tra apprendimento teorico ed esperienza pratica. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, desidero fare un ultimo passaggio in relazione alla riduzione del costo del lavoro: utilizziamo tutto il Fondo sociale europeo per abbattere il costo del lavoro, come fu autorizzato per la prima volta a fare il Governo Berlusconi con il credito d'imposta nel Mezzogiorno. Ne faremmo un uso semplice e certo negli esiti, certamente più efficace di tante politiche attive che hanno soddisfatto solo gli addetti ad esse. Viviamo un tempo nel quale la dimensione della crisi occupazionale è tale da sollecitare la ricerca di soluzioni pragmatiche e se necessario reversibili, orientate da risultati percepibili. È riducendo tasse e regole, come abbiamo sempre sperimentato, che si crea più lavoro. Con questi convincimenti, ribadiamo il voto favorevole del PdL.

voteremo a favore di questo decreto-legge, che non cancella il lavoro, senatore Uras, ma che prova a dargli una *chance* nelle condizioni date, date, tenendo insieme due temi fondamentali per garantire all'Italia di reggere una fase difficilissima, un cambiamento di sistema a cui la crisi economica ci sta traguardando. Abbiamo questo di fronte: una prospettiva di cambiamento sostanziale della qualità del nostro sistema produttivo e delle nostre relazioni sociali. Questa è la nostra sfida; una sfida che dobbiamo affrontare con determinazione, ma senza radicalismo, compiendo passi ponderati nella direzione del rafforzamento del sistema produttivo, della promozione e della tutela del lavoro, del sostegno alla ripresa dei consumi interni. L'accusa di moderatismo, di lentezza o di parzialità rivolta a questo decreto mal si sposa con la necessità di guadagnare un equilibrio nuovo, evitando scelte improvvise, svolte ideologiche e altri traumi, come quelli prodotti da scelte drastiche compiute nell'emergenza, nel corso dei due anni che abbiamo alle spalle. Alle condizioni date, nell'ambito di risorse modeste, soprattutto se raffrontate con la dimensione del problema che dobbiamo affrontare, il decreto indica una direzione di marcia, individuando un binomio fondamentale, che poggia sulla partecipazione al lavoro e sulla protezione del reddito la possibilità di risollevare l'Italia dalla grave crisi che la attraversa. Sul piano dell'accesso al lavoro, l'approccio «discriminato» del provvedimento risponde, oltre che a un orientamento imposto dalle regole di gestione dei fondi europei, con cui è finanziato, alla necessità di garantire sostegno alle fasce a maggior rischio di esclusione dall'esperienza lavorativa e dalla continuità della stessa. - e concordo con quanto già sottolineato dalla relatrice, senatrice Gatti - che proprio chi è più orientato alla protezione delle fasce più deboli critichi questo profilo del provvedimento.

Ma certamente l'alienazione totale dalla dimensione del lavoro di un'intera generazione, in vaste aree del Paese, così come l'esperienza del lavoro precario, scarsamente retribuito e scarsamente tutelato, è il fenomeno più preoccupante, perché prefigura la trasformazione strutturale Non è solo il rischio di impoverimento che ci preoccupa, ma la perdita dell'aspirazione all'autonomia e alla libertà che passa attraverso il lavoro, come elemento costitutivo del progetto di vita e trama della comunità civile e democratica. Un'esclusione che non colpisce tutti allo stesso modo: le giovani donne, i giovani al Sud, quelli con formazione insufficiente sono di fatto i più esclusi, ed è giusto che il provvedimento rivolga soprattutto a loro l'impegno a cambiarne le condizioni. Il profilo dell'attivazione al lavoro, il profilo dell'occupabilità è certamente quello più forte nella filosofia del decreto. Va in questa direzione soprattutto l'attuazione della cosiddetta garanzia giovani, oltre agli incentivi all'assunzione e alla trasformazione dei contratti

Questi ultimi agiscono, certo, nel facilitare le assunzioni attraverso un abbattimento, robusto per quanto transitorio, del costo del lavoro, ma non vi è dubbio che per affrontare in modo strutturale uno dei problemi uno dei problemi la via maestra sia quella della riduzione, per via fiscale, del cuneo abnorme che separa il reddito dal costo del lavoro. Obiettivo del Partito Democratico è cercare le condizioni per ridurlo progressivamente e strutturalmente con forme sostenibili e concrete, lontane da ogni provocazione e soprattutto da ogni demagogia: non si fanno promesse che non si possono mantenere nel tempo, non si raccontano bugie a chi è in una condizione già così precaria e distante dal lavoro! Gli incentivi avranno successo se, contestualmente, si opererà con determinazione alla ridefinizione del sistema di gestione delle politiche attive e passive del lavoro. Su questo esprimiamo un'opzione chiara: la cabina di regia tecnica, incardinata nella cosiddetta struttura di missione, rischia di non assolvere al compito urgente di ridisegnare in pochi mesi l'architettura e le funzionalità di un sistema pubblico, indispensabile per garantire programmazione e coordinamento dei livelli di servizio necessari per garantire, per l'appunto, le politiche attive e passive. Il nostro sistema pubblico è sottodimensionato, scarsamente integrato con quello privato e territorialmente disomogeneo: dobbiamo modificarlo in fretta, superando resistenze e veti incrociati o compiacimenti modellistici, per cercare, pragmaticamente, di realizzare rapidamente un disegno che cogliendo le peculiarità del nostro sistema formativo e produttivo lo sostenga nel cambiamento. In questa direzione va la nostra proposta di creare un'Agenzia a struttura federale, che speriamo trovi accoglienza in prossimi provvedimenti del Governo. Così come riponiamo molta fiducia nel fatto che le forme di flessibilizzazione del lavoro e la loro specificazione di settore trovino negli accordi fra le parti sociali che animano il lavoro la giusta dimensione, il giusto luogo per essere definiti. È questa l'aspettativa che riponiamo anche verso i confronti che si sono avviati intorno a Expo 2015: crediamo che essa sarà un'opportunità tanto più quanto all'interno del confronto sarà colto insieme

del lavoro di soggetti pienamente partecipi e rappresentativi. Voglio poi spendere qualche parola sul profilo di tutela sociale del decreto. L'innovazione della carta acquisti, affiancata alla preesistente *social card*, rappresenta una misura di lotta contro la povertà, in particolare quella minorile che in Italia colpisce il 20 per cento Non valgono su questo le polemiche, che purtroppo il Gruppo della Lega Nord continua a reiterare, sulla distribuzione territoriale delle risorse: le risorse devono essere impiegate dove con tutta evidenza il bisogno è maggiore e non facendo chi è più povero e chi ha più bisogno di misure per lo sviluppo! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non è incentivando la frammentazione del Paese e il divario territoriale che risolveremo il problema dello sviluppo che ci guarda tutti insieme: dalla crisi usciamo solo se il Paese è unito e ha un unico obiettivo. Abbiamo preso in quest'Aula un particolare impegno anche per aumentare la piena integrazione al lavoro delle persone con disabilità. Su questo c'è un *vulnus*, colleghi. La Corte di giustizia ci ha condannato per essere un Paese inadeguato a garantire parità dei diritti delle persone con disabilità. Avere introdotto con gli emendamenti misure in questo decreto che servono a superare questo *deficit* ci fa pensare di non aver lavorato per nulla. Che attraverso l'impegno nel sociale possa passare il processo di inclusione lavorativa dei giovani è testimoniato da molti emendamenti approvati, che promuovono l'occupazione attraverso l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, il recupero all'economia legale dei beni confiscati, il *tutoring* aziendale. Altro ruolo importante, e siamo contenti che questo sia avvenuto, ha il rifinanziamento del fondo nazionale per il servizio civile, su cui possono passare sia un miglioramento della partecipazione civile nel nostro Paese sia processi di attivazione al lavoro dei giovani. Per quanto attiene alle scelte in materia di fiscalità, il provvedimento opera un rinvio indispensabile non solo a traguardare una scadenza, che ignorata nei suoi effetti avrebbe prodotto un ulteriore insostenibile compressione dei consumi interni, ma anche a definire scelte adeguate e ponderate e una ridefinizione complessiva del profilo fiscale del nostro Paese. Abbiamo inoltre, questa mattina, finalmente dato approvazione a un emendamento su cui investivamo moltissime aspettative. Lo sblocco ulteriore del meccanismo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ci dà speranza di rimettere in marcia, anche attraverso questo strumento, l'economia. Gli impegni che il Governo ha preso per le prossime settimane rispetto alla definizione degli equilibri che devono caratterizzare alcune scelte fondamentali su IMU, IVA e ammortizzatori sociali dicono che dobbiamo, in questa fase, dare un segno del Paese che vogliamo. Vogliamo un Paese serio nel rispetto degli impegni e nella tenuta dei conti, in cui sul patto sociale fra lavoro e fiscalità si regge la convivenza e la democrazia. Il profilo fiscale che uscirà dalle prossime scelte deve garantire sostegno al lavoro e alla produzione, disegnando chiaramente una prospettiva di sostegno dei redditi e degli investimenti produttivi. Non possiamo permetterci, signor Presidente, nulla di diverso, non solo per ragioni di equità ma per necessità di crescita. Questo è l'impegno l'impegno che dobbiamo ai giovani, ai quali abbiamo dedicato il lavoro di questi giorni. È questo l'impegno che confido riusciremo a rispettare. vi sono numerosi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle che hanno chiesto di poter esprimere il proprio voto in dissenso da quello del Gruppo. Noi abbiamo esaurito i tempi. Anche i tempi degli interventi in dissenso sono stati oggetto del contingentamento, e i tempi sono stati largamente sforati

Non è possibile prevedere un contingentamento dei tempi sulla dichiarazione di voto in dissenso, in quanto quest'ultima può essere solo oggetto di valutazione dopo la dichiarazione di voto fatta dal Gruppo, che è

che regolamentano differentemente la discussione e la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto in dissenso può essere dichiarata al momento, in quanto può essere solo ed esclusivamente postuma

con i tempi contingentati e poiché, come ricordato, i tempi per il dissenso, che sono stati previsti e quantificati, sono stati utilizzati in maniera più ampia, anche per rispetto dei lavori dell'Assemblea,

alla dichiarazione di astensione espressa dal Gruppo in sede di dichiarazione di voto sulla legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013,

e poter portare avanti i lavori in maniera chiara e inequivocabile. Non ci basta la sua responsabilità. Noi abbiamo il diritto di andare avanti secondo il Regolamento, non secondo il suo senso di responsabilità.

Non ho tempo di esprimere il perché. Io rispondo a dei cittadini. PRESIDENTE. Lei deve annunciare il suo voto. Non è un'occasione in cui si può fare un intervento di merito. Dica all'Assemblea come intende votare in dissenso dal Gruppo. CASTALDI *(M5S)*. Non so se lei ricorda che qui ci hanno mandato nove milioni di cittadini italiani.

sulla base di questa situazione, convalidata poi dalla prima parte del comma 2 dell'articolo 109, lei ha sostanzialmente affermato che era terminato il tempo di pertinenza del Movimento 5 Stelle e che solo per ragioni di cortesia lei avrebbe consentito delle dichiarazioni di voto in dissenso secondo determinate modalità. Questo appartiene alla prassi del Senato. Ora, signor Presidente, con molta tranquillità le ragioni di cortesia che lei rivolge nei confronti del Movimento 5 Stelle esistono anche nei confronti del resto dell'Aula. E poiché a me non pare che la sua cortesia sia ripagata con analoga cortesia da parte del Movimento 5 Stelle la inviterei a procedere alla votazione.

Grazie.

Non posso ridare la stessa risposta sugli articoli 109 e 55 del Regolamento, che credo sia chiara.

con quest'intervento intendo dichiarare il mio voto in dissenso,

Invito i colleghi a non alimentare queste vicende. Prego, senatore Gaetti,

dell'articolo 84 del Regolamento: «I senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati

della discussione, ai senatori dissenzienti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza, un tempo determinato in aggiunta a quello attribuito a ciascun Gruppo». Quindi, i pronunciamenti sono numerosi ed ampi e stiamo andando ben oltre le limitazioni e le facoltà del Regolamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero prima di tutto esprimere la mia la mia solidarietà e quella del Gruppo del Popolo della Libertà, nonché l'apprezzamento a lei, signor Presidente, per come sta conducendo i nostri lavori.

Dico questo con molto rispetto per il vostro impegno politico, però ricordandovi che nella politica vi sono due dimensioni: c'è quella formale...*(Commenti

C'è una dimensione sostanziale, a cui noi tutti saremo

State dando una prova di maturità che è pari, anzi inferiore, a quella di molti consiglieri comunali. La questione sostanziale a cui noi tutti...

Presidente, sull'articolo 12 abbiamo notato una discrasia nella copertura di 150.000 euro, che abbiamo provveduto a correggere per esattezza.

particolare, pur dentro una cornice normativa di carattere generale, delle sorti dello stabilimento Ilva di Taranto. Con il primo decreto del 7 agosto dell'anno scorso, il Governo all'epoca ha inteso intervenire per fronteggiare la grave situazione ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, attuando il protocollo d'intesa tra Ministeri ed enti territoriali in cui erano previsti importanti interventi volti al risanamento ambientale dell'area di Taranto e alla riqualificazione produttiva ed infrastrutturale dell'area dello stabilimento Ilva.

Il 3 dicembre 2012, il Governo ha emanato un secondo decreto-legge, con il quale si introduceva il concetto di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, per i quali si potesse assicurare la continuità produttiva e la salvaguardia dell'occupazione, vincolandole alla piena attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Infine, siamo oggi ad un passaggio parlamentare decisivo per la trasformazione in legge del terzo decreto, sui cui contenuti si soffermerà in particolare il collega Bruni, con il quale innanzitutto si introduce la figura del commissario straordinario dell'impresa ritenuta di interesse strategico nazionale, la cui attività - recita il decreto - abbia comportato abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della reiterata inosservanza Basterebbe il richiamo ai ben tre decreti-legge, caso probabilmente unico nella storia industriale del nostro Paese dal dopoguerra, per dare il segno dell'eccezionalità di una vicenda, una vera e propria emergenza nazionale di straordinaria gravità, e non solo il dramma di una città che ha pagato un tributo altissimo a scelte industriali di un'altra Italia. Siamo, insomma, ad un passaggio cruciale, non solo per la vita dello stabilimento Ilva di Taranto, ma anche per l'intera storia industriale dei nostro Paese.

svolgendo dapprima una lunga visita allo stabilimento Ilva, accompagnati dal commissario, dottor Enrico Bondi, e dal subcommissario, professor Edo Ronchi, e poi incontrando in audizione le istituzioni locali e regionali, nonché i sindacati, le associazioni ambientaliste, l'ARPA Puglia e così via. Per chi lo vede la prima volta o per chi ci ritorna dopo molti anni, quello stabilimento dà sempre l'idea di un mostro d'acciaio che in tanti in questi ultimi anni hanno raccontato e rappresentato con sentimenti alterni e spesso contrapposti. Ciò che colpisce nel girarlo è innanzitutto l'enormità degli spazi, quel milione e mezzo di metri quadri (una volta e mezza la città di Taranto), in gran parte occupati da un immenso groviglio di tubazioni, di ferro e di nastri di cui si perdono alla vista l'inizio e la fine; poi i parchi minerari: 75 ettari in cui sono concentrati enormi cumuli di materiali, quali ferro e carbone allo stato pulviscolare, distanti poche decine di metri dal contiguo quartiere Tamburi.

l'arretramento di 80 metri dei cumuli dei parchi minerari, le centraline installate previste dall'AIA per il monitoraggio dell'aria, le coperture di una parte dei nastri trasportatori. insomma, di interventi importanti che hanno avviato il processo di mitigazione dei rischi di inquinamento dell'aria e del suolo, una delle condizioni per poter continuare l'attività produttiva, abbattendo in modo consistente gli inquinanti, prima ancora di avviare l'enorme opera di risanamento dei danni ambientali prodotti negli anni, vorrei dire nei decenni.

com'é stato possibile che questi interventi, del tutto ordinari e ormai presenti nella generalità degli stabilimenti industriali, all'Ilva siano stati realizzati solo negli ultimi mesi e solo dopo le vicende giudiziarie? Perché non dieci o anche solo cinque anni fa? Insomma, è difficile non avere la conferma che per anni, prima ancora che la magistratura intervenisse, prima che fosse predisposta un'AIA vincolante e stringente e prima che Governo e Parlamento agissero, insomma per troppi anni, quello stabilimento abbia prodotto a pieno regime, senza alcun rispetto di accorgimenti tecnici, impiantistici e di monitoraggio ormai largamente diffusi. È tutto qui il senso vero di questo provvedimento che ci apprestiamo ad esaminare e l'impegno gravoso che é dinnanzi al commissario straordinario e ai suoi collaboratori: realizzare i non più rinviabili investimenti tecnologici ed impiantistici per soddisfare le condizioni perché questo stabilimento possa continuare a produrre in sicurezza, abbattendo inquinanti e garantendo quella tutela della salute e dell'ambiente che la magistratura ha accertato non essere in linea con la normativa in materia, investimenti che per troppi anni l'Ilva ha negato o rinviato nel tempo. L'esame che ha svolto il Senato, sia nelle Commissioni riunite che nella importante missione a Taranto che ho richiamato, ci ha permesso di apprezzare i contenuti del decreto al nostro esame, non senza valutazioni critiche e unanimemente impegnati, tutti i Gruppi, voglio riconoscerlo, a migliorarne l'articolato per corrispondere quanto più efficacemente al grande sforzo che la vicenda reclama. Negli ultimi giorni è venuta dal Governo una forte preoccupazione, condivisa dalla maggioranza dei Gruppi del Senato, sui tempi di conversione in legge del decreto, alla luce dell'allungamento dei tempi di esame di altri provvedimenti, sia alla Camera che al Senato, che ha oggettivamente prodotto un pesante ingolfamento dei lavori parlamentari. Per queste ragioni, risultando pressoché impossibile immaginare la possibilità di una terza lettura del decreto Ilva alla Camera dei deputati entro il prossimo 3 agosto, abbiamo sposato l'orientamento ad un'approvazione definitiva in Senato, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Abbiamo inteso sostenere tale indicazione responsabilmente,

un provvedimento che contiene scelte decisive per la continuità produttiva dello stabilimento e per la sua ambientalizzazione. Non mancano punti su cui avremmo voluto contribuire ad un ulteriore affinamento del testo, a cominciare, tra l'altro - li richiamo velocemente - da una più puntuale definizione del ruolo del commissario, una valutazione delle funzioni di informazione e coinvolgimento delle comunità locali, finora assegnate al garante, i tempi di attuazione dell'AIA e dei correlati piani ambientale, industriale e sanitario, un più esplicito coinvolgimento delle agenzie ambientali, tempi e modalità di definizione del Piano strategico nazionale per la siderurgia. Su tali importanti questioni, con un ordine del giorno particolarmente puntuale che il Governo ha accolto, abbiamo impegnato l'Esecutivo, nelle Commissioni riunite, ad assumere iniziative conseguenti, da perseguire sia nell'ordinaria attività di monitoraggio dell'applicazione del decreto sia nell'adozione di alcune opportune ulteriori integrazioni di merito al testo di uno dei prossimi provvedimenti.

garantire con maggiore forza l'acquisizione di finanziamenti all'impresa funzionali alla predisposizione e all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del Piano industriale al commissario di sciogliere contratti con parti correlate del gruppo ritenuti incompatibili con tali piani; punti, questi, che noi riteniamo fondamentali per consentire davvero di concentrare tutte le risorse disponibili dell'impresa per le attività di risanamento ambientale. È poi necessario assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività del commissario straordinario la disposizione con cui lo stesso è impegnato a presentare una relazione semestrale ai Ministeri interessati e alle Commissioni parlamentari competenti, ivi comprese le iniziative di informazione e coinvolgimento delle comunità locali, compiti precedentemente affidati al garante.

di costante monitoraggio epidemiologico dell'area di Taranto, alla luce dei gravi danni alla salute riscontrati da varie fonti. Viene, infine, da questa complessa vicenda un'indicazione forte ad assumere il tema della valutazione dell'impatto sanitario dei grandi impianti industriali, su cui la Regione Puglia ha avviato una significativa iniziativa legislativa autonoma che ora merita e reclama un quadro nazionale certo, organico e coerente.

ma un pezzo decisivo del sistema industriale del nostro Paese e della nostra capacità di continuare ad essere un grande Paese manifatturiero, convinti, come siamo, che una moderna politica industriale non può non essere fondata che sulla sostenibilità dei processi produttivi, per uscire definitivamente dall'anacronistico dualismo lavoro-ambiente in termini finalmente positivi e costruire un futuro produttivo ed industriale in cui il vincolo, della sostenibilità sia davvero per il nostro Paese una grande occasione di crescita e sviluppo.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il decreto-legge n. 61 del 2013, oggi all'esame dell'Assemblea, come ha ricordato il senatore Tomaselli, è il terzo provvedimento d'urgenza emanato negli ultimi dieci mesi per far fronte all'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento Ilva di Taranto e delle aziende con le medesime caratteristiche e gli stessi problemi ambientali ed occupazionali. Prima di esso, infatti, il Governo Monti aveva prodotto il decreto-legge n. 129 del 2012, incentrato sulla necessità di risolvere la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di di interesse nazionale di Taranto, facendo seguito al protocollo d'intesa stipulato il 26 luglio 2012. Con tale protocollo erano, peraltro, stati stanziati 336 milioni di euro per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nel Comune di Taranto.

che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».

Infine, va segnalata - prima dell'adozione dell'odierno decreto - la pronuncia n. 85 del 2013 della Consulta, che ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del 2012, così come erano state poste dal GIP e dal tribunale di Taranto. Questo, in estrema sintesi, è l*'iter* dei vari provvedimenti intercorsi fino all'emanazione del decreto n. Con siffatto ultimo provvedimento il Governo ha introdotto modifiche significative, ulteriormente corrette nel passaggio alla Camera dei deputati. Il primo profilo da evidenziare riguarda l'applicabilità del decreto - e la relativa possibilità di decretare il commissariamento - ad ogni fattispecie di impresa di interesse strategico con esigenze concomitanti di tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro. Per determinare il carattere di «impresa di interesse strategico nazionale», secondo l'articolo 1, il requisito occupazionale minimo non può essere inferiore a 1.000 lavoratori subordinati; tale requisito, peraltro, è quello previsto nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ovvero nel decreto legislativo n. 270 del 1999. Altro requisito irrinunciabile per decidere il commissariamento è quello relativo all'attività produttiva dello stabilimento che comporti oggettivamente «pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute», a causa dell'inosservanza dell'AIA. Detta inosservanza, secondo il testo emendato alla Camera dei deputati, deve essere reiterata, implicitamente escludendo che una sola inosservanza dell'AIA sia sufficiente a determinare il commissariamento dell'impresa. Il commissario, per espletare la propria attività, si avvale poi di un subcommissario nominato dal Ministro dell'ambiente. Con il comma 1-*bis* la Camera dei deputati ha poi introdotto: l'obbligo nella procedura di commissariamento del parere delle Commissioni parlamentari;

L'ulteriore comma 1-*ter*, aggiunto dopo il passaggio del testo alla Camera dei deputati, consente di considerare il commissariamento quale deroga all'articolo 29-*decies* del codice dell'ambiente. Sempre all'articolo 1 si dispone

Degna di nota è la previsione dell'obbligo di informazione, da parte del commissario, sull'andamento della gestione dell'impresa; tale informazione va resa al rappresentante legale dell'impresa, al titolare ed al socio di maggioranza della stessa. In cosa consiste l'attività del commissario e del subcommissario, oltre all'esercizio della normale ed ordinaria attività d'impresa? Il *proprium* degli obblighi del commissario, alla stregua del presente decreto, consiste nella predisposizione di un piano industriale che, preceduta dalla redazione di un piano ambientale a cura di tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente (con competenze in materia di tutela ambientale, della salute e di ingegneria impiantistica), deve conformarsi a quest'ultima pianificazione. In altri termini, le attività di uno stabilimento di interesse strategico nazionale, una volta deciso il commissariamento, dovranno essere guidate da un piano ambientale, alle cui previsioni si dovrà adeguare ogni strategia industriale ed aziendale. Per essere ancora più espliciti: nel decreto si acquisisce la consapevolezza che il risanamento ambientale non può prescindere da un'accorta pianificazione aziendale e, nel contempo, si prende atto che ogni politica industriale di un'azienda commissariata, ai sensi del decreto-legge deve incentrarsi sull'obiettivo irrinunciabile della tutela ambientale e della salute. I due piani, quello ambientale e quello industriale, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione competente, il primo, e del Ministro dello sviluppo economico, il secondo. L'approvazione del piano ambientale, peraltro, vale quale modifica dell'AIA. Segue poi una disposizione relativa alla responsabilità del commissario, del subcommissario e del comitato di esperti, mutuata dall'articolo 6 della legge n. 231 per quanto attiene agli illeciti connessi all'attuazione dell'AIA e la previsione che il commissario non risponde delle diseconomie dei risultati *ex* articolo 2236 del codice civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave. Le somme eventualmente sequestrate per far fronte all'attuazione delle prescrizioni dell'AIA sono rese disponibili, dal giudice competente, al commissario per conseguire le predette finalità ed ottenere, quindi, la bonifica ed il risanamento ambientale. Infine, il Ministro dell'ambiente deve presentare ogni semestre una relazione sui controlli ambientali effettuati da ISPRA ed ARPA riguardo all'AIA rilasciata alle imprese, di cui alla fattispecie dei commi 1 e 1-*bis*. L'articolo 2 del decreto applica la fattispecie delineata dall'articolo 1 al caso di Ilva SpA, attribuisce poi agli ispettori ISPRA la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e fissa un termine di trenta giorni per la definizione, da parte del Ministro dell'ambiente, dei contenuti e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione per i procedimenti di cui all'articolo 29-*quattuordecies* del codice dell'ambiente. L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, prevede un contributo di 90.000 euro in favore del personale dell'ISPRA. Con l'articolo 2-*ter,* si escludono gli interventi di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, per 41,3 milioni di euro, Nel corso dell'esame in prima lettura è stata, poi, soppressa la figura del Garante introdotta dal decreto-legge n. 207 del 2012, attribuendo la dotazione economica di quest'ultimo al sostegno dell'attività dell'ISPRA. I compiti di informazione e consultazione espletati dal Garante vengono così affidati al commissario, che esercita gli stessi in accordo con Regione e altri enti locali.

A tal proposito, se volessimo nasconderci dietro il velo labile di una gratuita ipocrisia, oggi potremmo dire che tutte le complicazioni e le controindicazioni conseguenti al funzionamento dell'impianto industriale ionico ci dovrebbero far optare per una rapida chiusura dello stesso, magari rincarando la dose con un facile revisionismo delle politiche industriali dell'Italia degli anni Sessanta. Così continuando, potremmo poi censurare tutti gli stabilimenti industriali (le famose cattedrali nel deserto) realizzati nell'Italia del *boom*, con una logica dirigista che permeava di sé le strategie della Cassa del Mezzogiorno, evidenziando il fallimento o il cattivo funzionamento della gran parte di essi; ma si tratterebbe, appunto, di ipocrisia! La realtà è ben altra: nella città di Taranto Ilva è tuttora una realtà produttiva funzionante, che non può essere spenta in poche ore. L'esempio, più volte richiamato in questi giorni, di Bagnoli, di quell'area degradata, non bonificata, nonostante l'intervento *spot* della «città della scienza», è significativo: non si può chiudere una fabbrica con un giro di chiave per risolvere i problemi ultradecennali di degrado e inquinamento ambientale, mai affrontati seriamente prima d'ora. Gli esempi da seguire sono allora Nel corso della propria audizione il subcommissario Ronchi ha citato l'esempio dell'acciaieria Thyssenkrupp di Duisburg. Nella città tedesca, a ridosso dell'area urbana, sulla riva di un fiume vi è uno stabilimento della stessa capacità produttiva di quello di Taranto, che continua a svolgere la propria attività d'impresa strategica per il sistema industriale di quel Paese. Il decreto scommette proprio sulla possibilità di realizzare -anche in Italia - produzioni industriali, senza che ciò avvenga a danno della salute dei cittadini. Per ottenere tale obiettivo non si deve, però, concentrare ogni nostra attenzione solo sulle caratteristiche produttive e sull'ammodernamento degli impianti. Occorre ripartire anche da una più rigorosa ed omogenea attività di monitoraggio e controllo epidemiologico,

Concludo sottolineando che per giungere a decisioni condivise e appropriate occorrerà avere maggiori certezze sui dati epidemiologici e sulle valutazioni del danno sanitario. Ciò renderà più semplice il lavoro delle diverse autorità amministrative ed eviterà che ogni decisione su problemi così complessi sia riportata per l'ennesima volta nell'alveo patologico dell'indagine giudiziaria.

stenografico di seduta se non riesce a capire cosa si dice in Aula, e mi auguro che almeno riesca a comprendere le parole scritte. Non ho mai parlato di poteri deviati ma di forze esterne, né citato specifiche figure, che invece il senatore Esposito ama ripetere, probabilmente più per *slogan* elettorale che altro. Avrei parlato di magistratura inconsapevole e non colpevole, se il vice presidente Gasparri non mi avesse bruscamente interrotto, come invece gli piace fare solo con il Movimento 5 Stelle. Le prossime volte farò avere al senatore Esposito il testo completo di ogni mio intervento, in modo tale che possa dormire sonni tranquilli. Non entro nel merito della libertà di espressione altrui, proprio perché sono uno strenuo difensore della democrazia in ogni suo aspetto. Se mi è consentito, però vorrei leggere la parte di intervento che è stata tagliata anche dal Resoconto stenografico di Aula «Se mai arriverà in questa Aula il disegno di legge di ratifica dell'accordo internazionale italo francese del gennaio 2012, e voi colleghi lo approverete, sarete complici di una delle più grandi truffe perpetrate ai danni della collettività nazionale e delle finanze dello Stato. E su tutto questo, una unica regista, una regista che in passati processi sollevava la carenza di giurisdizione italiana ed ora senza scrupoli sfrutta una magistratura inconsapevole per i suoi perversi scopi. Colleghi, potete essere schiavi di questa società che fa il suo interesse privato? Non vedete che siamo ridotti a strumento inconsapevole per finalità molto distanti dalla nostra comunità? È ora di svegliarsi! È ora di dire basta! Vogliamo un sussulto di dignità!» Questo era quello che volevo dire per concludere l'intervento dell'altro giorno.

PAGLINI *(M5S)*. Uno vale uno, è un principio fondamentale su cui si fonda il Movimento 5 Stelle: uno vale uno quando ci sono proposte costruttive e voglia di partecipazione; uno vale uno quando si lotta per un'idea; uno vale uno è l'essenza stessa della democrazia. Nel mondo del lavoro è in atto un processo pesante e brutale di distruzione della persona, che viene sostituta dalla quantità di pluslavoro che riesce a fornire e che deve essere e che deve essere aumentata a dismisura, secondo i dettami del modello FIAT di Pomigliano o il *diktat* di Marchionne, distruggendo al contempo le tutele costruite dal dopoguerra ad oggi da due generazioni di lavoratori. Insufficiente ed inidonea risposta a questa situazione di crisi è stato l'accordo *ad* *excludendum* sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio, in cui si ribadiva il principio che attribuiva la titolarità negoziale solo ai sindacati con più voti. In un momento in cui è quanto mai necessaria un'azione unitaria a favore dei diritti dei lavoratori, la strada dell'esclusione non può portare vantaggi alla crescita e alla considerazione del lavoro in Italia. Uno vale uno è il principio che deve essere applicato anche alla tutela del lavoro. A luglio, la Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2013 è intervenuta in tema di rappresentanza sindacale dichiarando l'illegittimità dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. La Corte costituzionale ha giustamente evidenziato che si può dare risposta a queste esigenze attraverso una molteplicità di soluzioni e ha invitato il legislatore a intervenire. Il Parlamento deve dare una risposta alle richieste che vengono dalla Consulta. È necessaria una legge che precisi i criteri democratici, che consenta ai lavoratori, prima ancora che ai sindacati, di poter scegliere liberamente da chi e come essere rappresentati; una legge che garantisca la democrazia e la libertà e il diritto dei lavoratori in ogni luogo.

e non implementiamo la nostra nuova economia, la *green economy*, questi posti di lavoro non trovano poi ubicazione: possiamo agevolare quanto vogliamo, ma probabilmente a vuoto. Vorrei Vorrei porre all'attenzione il caso di un'azienda di Prato, la Wellness Innovation Project (WIP), produttrice di pannolini biodegradabili. In quest'Aula, già il senatore Panizza aveva parlato, ad esempio, di un'azienda dell'alta Italia che produceva lo stesso tipo di prodotto. prodotto. I prodotti di questa azienda pratese oltre ad essere apprezzati in tutta Europa, potrebbero rappresentare una soluzione importante per migliorare la gestione anche dei rifiuti,

questo non per motivi di mercato, non per assenza di un valido *business plan,* ma per mancanza del sostegno necessario, per mancanza di fiducia nel sistema Italia e quindi di disponibilità a spendersi e a rischiare in settori innovativi, per mancanza di normative chiare e incentivanti in un settore strategico e innovativo come la *green economy.* Forse la WIP di Prato verrà acquisita da imprenditori esteri e andrà a creare i 60 posti di lavoro previsti da qualche altra parte. Quindi, noi non stiamo perdendo soltanto il *made in Italy*, attuale ma anche il *made in Italy* del futuro. Dobbiamo ascoltare, dunque, chi ha idee per progettare un futuro diverso dando loro tutto il sostegno normativo necessario per uno sviluppo economico vero, a beneficio dell'ambiente. Sollecito quindi anche il Governo e il ministro Orlando ad attivarsi il prima possibile a tutela di questo settore produttivo e a rispondere quanto prima all'interrogazione del collega senatore Panizza.